senatore Sodano, non abbiamo né la certezza né la contezza del fatto che il Governo venga a riferire. Nel momento in cui dovesse esserci confermata la comunicazione del Governo e l'orario, allora potremmo organizzarci al riguardo.

ripercorrere quanto già avvenuto e di permettere ai senatori, che ovviamente lo ritengano opportuno, d'intervenire in Aula per esprimere la propria posizione in merito a questa questione che ha già interessato il Senato, questa Aula del Parlamento,

al di là di questa disputa regolamentare, se nel caso di dimissioni si applichi la norma del Regolamento per cui è previsto solo un intervento per Gruppo, oppure come in parte avvenuto nel caso delle dimissioni del senatore Malabarba, trattandosi financo, in molti casi, di valutazioni politiche che attengono alla persona, per capirci, non disciplinate dall'agire del Gruppo, a nostro avviso, ogni senatore dovrebbe poter esprimere un'opinione in merito alle dimissioni. Tuttavia, rimandando a un chiarimento in materia, vorrei richiamare due questioni, riferendomi al dibattito che si è svolto la scorsa settimana quando si è discusso delle dimissioni del senatore Malabarba e delle dimissioni, poi respinte dall'Assemblea della senatrice Livia Turco. In primo luogo, io sono un parlamentare da poco eletto, tuttavia, mi sono documentato, ho letto, ho studiato: c'è un'antica prassi parlamentare per la quale, per la verità, in prima istanza, le dimissioni venivano quasi sempre - sottolineo il quasi - respinte, per un segnale di solidarietà, di attenzione e di stima verso l'onorevole o senatore

chi, come me, è espressione di una forza politica e ha anche una storia di militanza di cui è orgoglioso, sa bene che una cosa è il mandato parlamentare e una cosa l'appartenenza ad un Gruppo. vorrei con pacatezza chiedere ai senatori - mi rendo conto che il momento è particolare - come mai potremo costringere un senatore a rimanere senatore quando eventualmente l'Aula gli negasse le dimissioni. Questo principio, per la verità, sul piano umano e sostanziale è stato accettato per il senatore Malabarba:

il fatto che oggi questi senatori che chiedono di dimettersi siano membri del Governo: questo può essere l'argomento - perché come tale è stato addotto - per il quale l'opposizione teorizza una volontà di

dell'economia, deve prima chiarire questo equivoco. Ma per favore, se noi sancissimo questo meccanismo, seppure legati alla contingenza, allo scontro politico, sanciremmo un principio per il quale la libertà del parlamentare è messa in discussione. Colleghi senatori, per carità, mi rendo conto che lo scontro politico fa dire una cosa e il suo contrario, ma abbiamo almeno il coraggio di dire: «Noi non voteremo le dimissioni perché vogliamo crearvi un danno politico, perché vogliamo fare in modo che i Sottosegretari siano sempre in Aula, che i Ministri siano sempre in Aula in Aula e, visto che c'è una maggioranza risicata, vi vogliamo creare problemi nell'azione di Governo». Infine, l'idea che il Parlamento controlli il Governo attraverso la presenza di Ministri e di Sottosegretari senatori mi sembra una follia, il ruolo d'indirizzo nei confronti del Governo, il ruolo di controllo attraverso gli atti ispettivi

membri della Camera o del Senato; altrimenti, francamente questa discussione è stucchevole. Ecco perché invito l'Aula a dichiarare un orientamento favorevole all'accoglimento delle dimissioni dei senatori che le hanno presentate e credo che bisogna evitare che l'acuirsi dello scontro politico metta in discussione un principio di fondo: il parlamentare liberamente esprime i propri elettori, non ha un vincolo di mandato rispetto al partito e nessuno, ma proprio nessuno, potrà obbligare una parlamentare o un parlamentare a continuare ad essere parlamentare se non lo vuole, né questo può essere un elemento di ricatto politico, come per esempio è avvenuto nei confronti del senatore Malabarba, che ha dovuto ritardare di oltre un mese le sue dimissioni, con seri problemi personali, perché la contingenza politica non ha consentito di trovare una convergenza perché quelle dimissioni fossero accolte. Vi prego di discutere e di riflettere. Chiedo che vengano accolte le dimissioni dei senatori che le hanno presentate.

fa ostruzionismo, il Governo chiede il voto di fiducia. In questo caso assistiamo all'ostruzionismo

Tecce, non perché siamo più bravi, ma perché purtroppo abbiamo più anni di lei, siamo in Parlamento da tanto tempo. Fino al 1980

Le dimissioni presentate quest'oggi hanno a che fare con una scelta di carattere politico che non possiamo assolutamente accettare.

Quando vi saranno le dimissioni di tutti i Ministri e di tutti i Sottosegretari che fanno parte del Governo, il Gruppo di Alleanza Nazionale potrà rivedere la sua posizione. Finché si manterrà questa situazione, però, continueremo a votare contro. Desidero aggiungere che un collega senatore ha rilasciato oggi una dichiarazione che non riguarda l'argomento, ma quanto accaduto questa mattina. Il senatore Salvi ha dichiarato: «In un contesto così complesso e difficile come il Senato non si può agire con questa dose di dilettantismo». E conclude la sua

prenda contezza di questo e si ritirino definitivamente la dimissioni.

è stato accennato da alcuni autorevoli colleghi, esso investe i rapporti tra Governo e Parlamento; indirettamente, investe la natura parlamentare della nostra forma di Governo; il tema, addirittura, giunge ad investire la questione del rapporto fiduciario che, all'interno di una forma di Governo parlamentare, lega il Governo al Parlamento. questioni molto rilevanti, tutte le soluzioni sono possibili e, detto con franchezza, abbiamo sentito opinioni, per la verità, alquanto singolari. Anche all'interno delle forme di Governo parlamentari, nel mondo, esistono soluzioni che prevedono,

di Governi che sono rimasti rigidamente all'interno della forma di Governo parlamentare e che hanno previsto un'ampia presenza al loro interno di persone che non ricoprivano una carica parlamentare.

di Governo e come immaginiamo che essa debba evolvere nella prassi. Possibilmente, personalmente ritengo che prima o poi dovrà cambiare, anche grazie a riforme adeguate. Purtroppo, come spesso capita nelle Aule parlamentari, arriviamo a questa discussione molto male,

una forzatura, un utilizzo piuttosto spregiudicato - i colleghi lascino che lo dica - della prassi secondo la quale le dimissioni dei membri del Parlamento almeno una prima volta vengono respinte, come attestato di stima e atto di cortesia

per indebolire la capacità della maggioranza di essere stabile e consistente, di realizzare l'indirizzo politico sulla base del quale quella maggioranza ha ricevuto il consenso da parte degli italiani.

avviene noi, attraverso un *escamotage* tecnico, tenteremmo di sovvertire la maggioranza nel Senato quale è stata determinata dal libero voto degli italiani.

non già a rendere più efficaci i lavori di questo ramo del Parlamento (in quanto non ritengo che il ruolo dell'opposizione sia di rendere inefficaci i lavori del Parlamento

possa condurre a compimento le misure, le leggi, le proposte di legge necessarie ad attuare quell'indirizzo politico in base al quale è stato scelto dagli elettori attraverso

la sua opinione è autorevole rispetto alla questione che intendo porre, che è riferita all'articolo 55 del nostro Regolamento, che disciplina le modalità della discussione in Aula. Lo spunto me lo offre l'intervento svolto poc'anzi dal senatore D'Amico, il quale è arrivato a teorizzare che, siccome gli italiani hanno votato, l'appuntamento è cinque anni dopo e non ogni giorno nelle Aule del Parlamento, per cui l'opposizione, se la maggioranza non ha senatori, sostanzialmente dovrebbe rinunciare a far entrare in Aula i propri senatori. È un argomento piuttosto bizzarro,

senatore D'Amico e quanti come lui stanno praticando in queste ore l'ostruzionismo di maggioranza - che, come ha detto il presidente Matteoli, è legittimo: la differenza è che noi non possiamo contare sul voto di fiducia, mentre voi sì dimenticano che questa mattina sono mancati non 11, ma 13 senatori della maggioranza, visto che mi rifiuto di pensare che i senatori a vita siano membri della maggioranza. numero di 13 senatori è l'equivalente (e più) di un Gruppo parlamentare, per questo abbiamo parlato di problema politico legato alla sconfitta della maggioranza sul decreto in materia di sfratti, su cui avete inscenato una polemica incredibile, per il semplice motivo che gli sfrattati non subiranno conseguenze, perché non avrebbero avuto effetti benefici dall'approvazione di un decreto senza copertura finanziaria. In sostanza, siete stati innervositi dal fatto che l'unico sfrattato che rischia davvero qualcosa si chiama Romano Prodi.

Voglio sapere se siamo in sede di discussione generale, che non esiste sull'istituto delle dimissioni, o se siamo in sede di dichiarazione di voto che credo, per lettura attenta del Regolamento, sia consentita ad ogni senatore ed è la prassi che si sta introducendo oggi. oggi. Voglio sapere dal Presidente del Senato, visto che la materia non è tra quelle contingentabili, per il futuro, perché la si può scampare per queste dimissioni, casualmente, se mobilitate proprio tutti, potrebbero anche passare, ma per il futuro, quando toccherà a ciascuno di tutti gli altri, lei sappia Presidente che oggi si sta stabilendo il precedente per cui tutti ci possiamo iscrivere a parlare ogni volta che si vota su dimissioni e siccome sono dimissioni per motivi politici, ci sentiremo tutti legittimati ad intervenire per motivi politici il giorno in cui ci dovessimo accorgere che i numeri sono favorevoli all'Unione è non a noi. Infatti, se questa è la regola, dobbiamo intenderci che è una regola che vale anche per il futuro.

io dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani sulle dimissioni del senatore Pinza. Cercherò di svolgere un ragionamento per tentare di convincere i rappresentanti dell'opposizione della necessità di accogliere tali dimissioni.

Credo che l'opposizione stia facendo giustamente il suo mestiere; del resto, sia il presidente Matteoli che il senatore Storace hanno ripetutamente dichiarato che ci troviamo di fronte a dimissioni politiche che devono essere valutate in termini politici e dunque in termini politici i Gruppi parlamentari si devono confrontare per esprimere l'orientamento sulle dimissioni

credo inoltre che sarebbe opportuno tentare di svolgere un ragionamento più generale circa la compatibilità di questa scelta politica assunta dall'opposizione a causa della necessità, per l'opposizione stessa ovviamente, di mettere in crisi il Governo nel suo rapporto con la maggioranza e, invece, la necessità di pensare in generale agli interessi del Paese.

Mi spiace dirlo, ma questo è ciò che si verifica in questo ramo del Parlamento e questo gruppetto consistente ha un comportamento reiterato. Infatti, si è verificato più volte che le dimissioni non siano state accolte grazie anche al comportamento di alcuni senatori che, ovviamente, fanno parte della maggioranza. Pongo questo problema, Presidente, perché è un problema che abbiamo noi nei confronti del Governo; è un problema che questa maggioranza deve risolvere in qualche modo. Il problema, allora, è il funzionamento

Sappiamo qual è la risposta dell'opposizione: nessuno ha obbligato i senatori dimissionari ad assumere cariche di Governo e, quindi, adesso la maggioranza si deve fare carico di tale responsabilità.

che sottopone le istituzioni a questo balletto inverecondo, dove volta per volta non si capisce bene quale sarà il risultato delle votazioni. Una legge elettorale che ha tolto ai cittadini elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, ma ha assegnato tale responsabilità alle segreterie dei partiti. E il Parlamento, le istituzioni sono costrette a subire le conseguenze di una legge elettorale Attraverso la presenza nelle istituzioni, attraverso la scelta dei candidati a Ministro o a Sottosegretario, il Parlamento, grazie a questa legge elettorale sbagliata, ha la possibilità di determinare scelte che poi devono essere

Il Parlamento eletto attraverso questa legge elettorale sbagliata ha la possibilità di determinare il cambiamento rispetto ai propri rappresentanti. Credo che questo sia un problema generale, che va posto, e che la questione dovrebbe essere

le modifiche da apportare alla legge elettorale, che ci consentano di non sottoporre le istituzioni - come dicevo prima - a questo balletto inverecondo. Detto questo, non è che ritenga che,

del Paese e il funzionamento delle istituzioni, verrebbe assegnato al partito che prende più voti e, quindi, se ne cambia natura, se ne cambia la finalità, che era appunto quella di garantire la possibilità che le istituzioni funzionassero e che vi fosse una maggioranza per garantire la governabilità al Paese. Credo che, da questo punto di vista, dovrebbe essere colta, da parte di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, attraverso il voto di accettazione delle dimissioni, aprire una fase nuova di confronto sulla legge elettorale, per modificarla e renderla più corrispondente alle necessità del Paese. *(Applausi

chiari, interni a questa Camera in particolare, cioè al Senato. Sono una di quelle persone che ritiene che non si debbano avere doppi incarichi; questo può apparire in contraddizione con quello che andrò dicendo. È altrettanto vero,

quindi trovata una modalità comune, che vorrebbe dire anche rimettere in discussione e ripartire sulla legge elettorale. Ma questo viene dopo. Oggi il Parlamento è quello che è stato eletto attraverso la legge elettorale elettorale che vige tutt'oggi; questo rimane il primo problema. Naturalmente non vi è niente di personale nei confronti dei Sottosegretari e dei Ministri che chiedono di fare solo e unicamente il lavoro per il quale sono stati scelti, ossia quello di Governo, e non tanto di stare al mandato elettorale; un mandato che comunque è stato ricevuto dai cittadini. È evidente che questa è una contraddizione all'interno della democrazia: non si riesce a capire per quale ragione, da un lato, devono essere date le dimissioni e, dall'altro lato, perché queste persone si devono dimettere. Non sto rincorrendo me stesso per tentare di trovare una soluzione; ma, personalmente, non posso ritenermi d'accordo su questo. Quindi, in realtà, credo che aspetterò tutto il dibattito e sentirò le altre persone che ritengono di intervenire su questo tema. Mi pare che all'interno del nostro stesso Gruppo, caro senatore Ripamonti, vi sia una dissidenza su questo tema che non riguarda solo il sottoscritto, ma anche altre persone;

decreto sugli sfratti, cioè uno degli interventi che più aspettava il Paese, anche perché riguarda milioni di cittadini; tale questione è stata affrontata in maniera probabilmente sbagliata da parte dalla maggioranza, oggi divenuta minoranza all'interno dell'Aula. Vi è un dato politico in questo. Francamente credo che andasse colta la richiesta di sospendere i lavori avanzata anche da parte dell'opposizione. Dico questo perché, nel momento stesso in cui non si è riusciti ad espletare il nostro mandato su una questione come quella... *(Proteste dal

ci richiamiamo, però, alla Presidenza. Come ha detto opportunamente il collega Storace poc'anzi, la Presidenza sta instaurando ed avvalorando un principio secondo il quale, al di là del rispetto formale del Regolamento, il quale prevede che, in presenza di dimissioni da votare,

se gli interventi in dissenso saranno identici a quelli del collega che ci ha preceduto, ci accingiamo evidentemente a votare in Senato forse in piena notte: ne prendiamo atto, Presidente. Le regole peròvalgono per tutti

a tempi molto, molto ristretti e addirittura a volte Presidenze che hanno preceduto la sua, presidente Marini, anche del presidente Mancino, hanno invitato i colleghi che esprimevano il voto in dissenso a farlo pervenire addirittura ai banchi della stessa Presidenza. Comunque, attendiamo da lei una risposta, così come le significhiamo che è intenzione di questa coalizione arrivare in ogni caso ad un voto prima di qualunque sospensione dei lavori d'Assemblea, così come da lei anticipato. *(**Applausi dal

della collega chiedere che si votino queste reiterate dimissioni. Veramente eravamo convinti che, esistendo un problema politico interno al centro-sinistra su queste dimissioni, lo stesso centro-sinistra avesse fatto mente locale circa l'inopportunità di questo percorso, in particolar modo all'indomani del voto negativo sulle dimissioni della senatrice Turco. In ogni caso, signor Presidente, siamo vigili su quanto sta accadendo oggi pomeriggio in Aula. Siamo pronti a fare anche le ore notturne pur di arrivare ad un voto, ripeto, prima di qualunque sospensione dei lavori ed abbiamo preso atto anche di un cambiamento di idee del Governo. abbiamo ascoltato con attenzione l'intervento del rappresentante del Governo e la sua disponibilità a venire a riferire domani sui fatti che si sono verificati oggi. Apprendiamo, invece, di un cambiamento di programma: il Governo viene oggi pomeriggio, anziché domattina.

Presidente, non ho mai messo in dubbio la sua correttezza nel gestire l'Assemblea. So come lei è fatto, non soltanto da quando è Presidente del Senato, ma per una vecchia conoscenza. Quando il senatore Storace, non nel suo intervento ma rispondendo a dei colleghi della maggioranza, oggi opposizione,

Signor Presidente, credo che l'interpretazione da lei data dell'articolo 109 del Regolamento sia assolutamente inappuntabile. Essa infatti non soltanto corrisponde al testo della norma e, come si suol dire, *in claris non fit interpretatio*, ma trova conferma in una prassi costante. Vorrei ricordare ai colleghi che, quando si procede al contingentamento del voto su un provvedimento, si attribuisce uno specifico spazio ai senatori che si esprimono in dissenso con un eccesso di restringimento, ma questo tema lo potremo approfondire in altra sede), perché anche i senatori dissenzienti devono avere un minimo di tempo per poter esprimere il loro punto di vista.

Semmai il quesito che dobbiamo porci è se su questo tipo di votazioni siano ammissibili dichiarazioni a nome dei Gruppi, ma ciò porterebbe a dire che tutti i senatori, non soltanto meno della metà del Gruppo, possono esprimere il loro voto. Mi sembra, quindi, signor Presidente, che la sua decisione sia assolutamente ineccepibile e che tutti i senatori in dissenso con le posizioni espresse dai rispettivi Presidenti fino alla concorrenza della metà meno uno dei membri del Gruppo stesso, abbiano il diritto di intervenire in sede di dichiarazione di voto e per dieci minuti.

sono state sollevate dai Capigruppo dell'opposizione due questioni che onestamente ritengo serie. è quella sollevata dal presidente Matteoli, che è stata egregiamente ripresa dal collega Salvi. Signor Presidente, il problema esiste:

ogni collega abbia il diritto di parlare e di dichiarare il proprio voto. È altrettanto evidente che i colleghi che dissentono hanno il diritto di esprimere il loro dissenso. Il presidente Matteoli

esperto di rappresentanza della maggioranza parlamentare, ci ha garbatamente esortato

che abbiamo per la Presidenza, è una questione che va oltre la semplice applicazione del Regolamento; occorrerebbe pertanto una vera e propria interpretazione per capire se, in presenza di un voto segreto,

però, è interesse anche dell'opposizione, credo, per il futuro (se essa aspira prima o poi, mi auguro più poi che prima, a diventare maggioranza), ad evitare precedenti negativi. La Conferenza dei Capigruppo è allora nella quale la ragionevolezza può far trovare ai vertici istituzionali dell'Assemblea un *modus* *procedendi* in grado di evitare la nascita di precedenti negativi. Signor Presidente, la questione

dei Capigruppo. Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo, penso che i vertici istituzionali dell'Assemblea debbano affrontare il nodo stamattina l'ho definito politico, per certi versi, perché tale è - di un situazione contingente che si è creata. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito; per i motivi che ho detto (alcune assenze per malattia, altre per missioni), c'è una situazione d'Aula atipica, nel senso che la maggioranza per queste circostanze ha uno, due, tre voti in meno dell'opposizione. Questo fatto, Presidente, non può costituire uno stravolgimento della vita dell'Assemblea in maniera permanente e strutturale e determinare una serie di voti a catena che stravolgono i rapporti di forza. Sono situazioni che possono capitare,

possa affrontare questa situazione e questa circostanza e deciderne la gestione in modo ragionevole e nell'interesse delle istituzioni. *(Commenti

solito. Siamo di fronte ad una discussione di carattere regolamentare che non può essere risolta in punta di Regolamento, come si dice, perché il vero problema che abbiamo davanti è quello di una maggioranza che strumentalizza apertamente il Regolamento per impedire all'opposizione di pronunziarsi politicamente su di un argomento regolarmente programmato. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).* Allora, più che fare un richiamo al Regolamento, mi consenta, signor Presidente, di fare un appello a lei perché, nell'ambito dei suoi poteri, garantisca all'opposizione il diritto di esprimersi compiutamente

Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei motivare perché voterò contro le dimissioni del senatore Pinza. Parto da una considerazione: sono favorevole al principio generale che chi svolge funzioni di Governo non deve svolgere anche funzioni parlamentari. Devo dire che nei consigli comunali questo principio è stato pienamente attuato e ha perfettamente funzionato: chi è consigliere non è assessore e chi è consigliere e diventa assessore automaticamente viene dimesso senza votazione, ma per un'incompatibilità precisa, stabilita sulla base di norme, regolamenti e statuti comunali. Perché sono favorevole a questo principio? Perché offre la possibilità di aprire maggiori spazi d'impegno alla politica, vi è un enorme bisogno di rinnovamento, di dare spazio a giovani, a donne, a nuove competenze per nuove sfide che ci attendono su tanti temi. È chiaro che la sovrapposizione tra incarichi parlamentari e incarichi di Governo deprime queste opportunità, non soltanto in questa legislatura (è evidente, i numeri risicati della maggioranza rendono ancora più complessa la gestione quotidiana di quest'Aula), ma anche in tutta la precedente legislatura legislatura i Sottosegretari o i Vice Ministri non hanno mai partecipato, almeno nella mia Commissione, ai lavori, proprio perché impossibilitati, dovendo seguire attività di Governo esterne o interne alle Aule parlamentari, a dare un proprio contributo in quanto parlamentari eletti dal territorio. Ovviamente, non c'è nulla di personale nei confronti della legittima richiesta del senatore Pinza di vedere accolte, con la loro presentazione, le dimissioni da quest'Aula del Senato, ma penso che vi sia un altro modo di risolvere il problema: che vengano affidati incarichi di Governo soltanto a soggetti esterni al Parlamento e che questo venga stabilito come una regola che dovremmo discutere in senso generale e adottare come codice di comportamento all'interno dell'Unione. Altrimenti, come sta accadendo oggi, si entra nel campo della discrezionalità tra chi si dimette e chi non si dimette; si entra, tra l'altro, in quella difficilissima questione non risolta delle dimissioni che non sono poste in capo ai singoli, perché in realtà le dimissioni dei singoli, senatori o deputati, sono nella disponibilità dell'Aula, come stiamo verificando anche oggi. Esse quindi si prestano a una straordinaria battaglia politica da parte del centro-sinistra, che legittimamente chiede (con il senatore Pinza, in questo caso) che si possa abbandonare il seggio senatoriale per potersi meglio dedicare ai lavori di competenza del proprio Dicastero;

quest'Aula - come una battaglia politica per mettere in difficoltà una maggioranza risicata di centro-sinistra. Non ritengo che questo sia lo strumento più opportuno per arrivare a delle considerazioni generali di opportunità politica su una regola che dovrebbe valere in termini generali per tutti, senza che sia rimessa alla disponibilità, come oggi, Tra l'altro, ricordo che il senatore Pinza ha già presentato le sue dimissioni e almeno una volta l'Aula le ha respinte. Queste sono le ragioni specifiche che mi inducono a votare diversamente dal mio Gruppo, quindi non ragioni ragioni personali. Ovviamente comprendo le necessità da parte del senatore Pinza di reiterare le proprie dimissioni, ma credo che dovremmo spostare questa riflessione non tanto sui casi singoli, ma su una regola generale che stabilisca una precisa incompatibilità tra incarichi di Governo e incarichi parlamentari. Queste sono i motivi che mi inducono a dissentire dal mio Gruppo, il quale voterà a favore delle dimissioni, proprio per accogliere la richiesta del senatore Pinza. Credo però che questa sarebbe una sorta di scorciatoia per non affrontare un problema generale, che è quello di come allargare gli spazi della politica, in particolare quelli legati agli incarichi di Governo, che richiedono passione, tempo, competenza e che, se vogliono essere vissuti pienamente, sono incompatibili con quella rappresentanza territoriale che i cittadini, pur con questa orrenda legge elettorale che non ha neanche assicurato loro di poter esprimere preferenze, ci hanno invece demandato in quest'Aula legislativa.

anche se contrasta con la volontà espressa dal singolo (e non so fino a che punto questo sia legittimo). Per il gioco della battaglia parlamentare, è legittimo che le opposizioni respingano le dimissioni, creando difficoltà alla maggioranza,

Prodi - anticipata anche in campagna elettorale - di chiedere a tutti i deputati e i senatori che avessero assunto ruoli nell'Esecutivo di rassegnare le dimissioni sia stata una scelta giusta e sarei per condividerla.

anche per problemi interni alla maggioranza. Ho sofferto molto anche per le vicende del mio amico Malabarba, che ha chiesto di potersi dimettere per motivi assolutamente personali.

abbia ragione la senatrice Donati quando dice che su questa materia sarà bene che si provveda in modo da evitare il verificarsi di certe situazioni. Io sono assolutamente per l'incompatibilità. Non voterò a favore delle dimissioni per vedere annullato il mio voto e, ancora una volta, per mettere coloro che sono disponibili a reiterare le proprie dimissioni nelle condizioni di fare - come si dice al mio paese - una figuraccia.

In questo Paese c'è gente che fa il Presidente del Consiglio, l'onorevole, il presidente di vari consigli di amministrazione, persone con

a rinunciarvi per svolgere appieno il loro ruolo di rappresentanza in modo che anche questa Camera, che ha una maggioranza risicata, non sia tutti i giorni ostaggio

vedersi accettare delle dimissioni bisogna contrattare. Infatti, non vi sono mica solo i sacri principi dell'opposizione, c'è anche il vil denaro, che alla fine fa parte dello scambio di voti.

perché le dichiarazioni di voto non sono vuote parole, ma un preciso impegno che i Capigruppo - o chi parla a nome del Gruppo - prende a nome di tutto il Gruppo, oppure sono un preciso impegno del singolo senatore. Pertanto, dovrebbe accadere - e dovrebbe essere una preoccupazione della Presidenza - che, conseguentemente, il voto sia coerente con la dichiarazione: credo che questo sia un dato assolutamente incontrovertibile.

perché nel momento in cui dichiaro personalmente cosa voterò, derogo dal voto segreto. Se il voto è indisponibile perché deve, in qualche modo, tutelare la libera volontà del senatore, ciò non è possibile.

l'impressione che la Presidenza abbia interpretato l'articolo 109 del Regolamento in questo senso, avendo ammesso le dichiarazioni di voto personali. Se questo è vero, deve essere incontrovertibilmente vero il fatto che nel momento in cui il senatore dichiara *urbi et orbi* il proprio voto, egli rinuncia

qualcos'altro. Signor Presidente, la prego di chiedere al senatore Tibaldi di chiarire bene questo concetto perché noi non abbiamo barattato niente con nessuno! Poiché siamo in un'Aula parlamentare,

ha chiesto un determinato incarico in una Commissione, che quell'incarico non poteva essere assegnato

Voglio dire al senatore Tibaldi che tra i Gruppi la discussione, specialmente in uno schieramento e nell'altro, dell'assegnazione delle posizioni nelle varie Commissioni è un fatto quotidiano per tutti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho vissuto una vita di dissidente e ho cercato di essere un po' l'angolo che sporge,

un lavoro serio in riferimento agli atti governativi e alla presenza in quest'Aula, che, come si sa, ha i numeri risicati. Ricordo che già da tempo ripeto che le mancate dimissioni dei senatori con incarichi governativi pongono e sono un problema politico più serio di qualsiasi discussione sull'Afghanistan. In realtà, ha ragione l'opposizione, quando dice che sono dimissioni politiche. E le ragioni sono molto differenti dalle motivazioni personali, che tutti abbiamo accolto per umanità, per necessità e perché c'è anche un diritto e un dovere alle dimissioni, e dalle dimissioni precedenti. In questo caso, in effetti, si sollevano i problemi che attengono alla democrazia, alla rappresentanza e a cosa si intenda per rappresentanza, nonché il problema degli incarichi, della loro compatibilità tra legislativo

la Grecia, già allora escludeva i barbari, le donne e gli animali dalla *polis*, dalla democrazia e l'urlo di Antigone già diceva di quanto le donne, la soggettività delle donne e il loro sapere fosse comunque al di fuori della cittadella del potere. caso però ci troviamo di fronte ad una crisi che è data, da una parte, del sistema integrato delle comunicazioni di massa, e quindi dalla impossibilità di governo della complessità da parte dell'utente di fronte alla partecipazione, e, dall'altra, ci troviamo di fronte proprio alla crisi della individualità, nell'anonimato delle nostre città, nella incapacità di relazioni e specialmente nella incapacità di conoscere e quindi decidere. Che cosa c'entra tutto questo con la questione delle dimissioni? C'entra molto, e la domanda che già la senatrice Anna Donati poneva sulla possibilità di incompatibilità non era, a questo punto, solo una necessità per la maggioranza di disporre di soggetti in carne ed ossa,

del modo in cui siamo eletti. Infatti, vogliamocelo dire, con l'ultima riforma elettorale - ma secondo me anche con quelle precedenti - il potere decisionale su chi veniva eletto era ormai nelle strutture

l'adesione e l'elezione della rappresentanza salta; salta nella rappresentanza verso i collegi - tra l'altro io questo l'ho trovato sempre giusto perché chi siede qui rappresenta il popolo italiano

patto di lealtà tra gentiluomini sulle dimissioni - che anche le dichiarazioni sulle sue presunte dimissioni darebbero a tutta l'Italia la sensazione che il Governo duri. Signor Presidente, colleghi senatori, ci troviamo a votare la richiesta di dimissioni di due colleghi. Non è la prima volta: in una precedente occasione molti colleghi hanno notato che, non per caso, il voto in queste circostanze è obbligatoriamente segreto. È stato letto nella norma regolamentare un invito che il nostro Regolamento implicitamente ci rivolge a non politicizzare questo momento e a dare un grande spazio alla libertà di coscienza di ogni componente dell'Assemblea. Ad ogni buon conto, dunque, inviterei l'opposizione a non strumentalizzare tale dibattito, dato che riguarda questioni non strettamente politiche, come si vorrebbe far pensare, ma un problema di ordine istituzionale e costituzionale costituzionale che ha una grande rilevanza: quello del rapporto tra i poteri, il rapporto che deve vigere tra il Parlamento e l'Esecutivo. Dal mio punto di vista, ritengo che tali problematiche di ordine costituzionale necessitino di essere approfondite in altra sede anche con più tempo a disposizione. è necessario occuparsi della risoluzione di un problema concreto che è quello dell'impossibilità, per alcuni colleghi, di svolgere contemporaneamente le impegnative funzioni di senatore e portare avanti le altrettanto impegnative attività di Governo. Queste sono le ragioni e le motivazioni che dovrebbero spingere all'accoglimento delle dimissioni dei componenti del Governo: mi riferisco alle dimissioni del collega senatore Bubbico e del senatore Pinza. L'opposizione le rifiuta solo per strumentalità politica, nella speranza di danneggiare in questo modo la maggioranza, essendo noto tutti che la stessa maggioranza, in questo ramo del Parlamento, è di poche unità di voto. È la maggioranza, sì; la maggioranza c'è: è coesa, è compatta; episodici e rari momenti di *défaillance* non ne compromettono la stabilità.

dopo le tante discussioni e disquisizioni avvenute in quest'Aula, ho avuto paura di compromettere quel sostegno che volevo accordargli. Ecco, non vorrei incorrere in questo stesso errore. Tutto ciò accade proprio perché abbiamo ingoiato un sistema elettorale, anzi, una stortura di sistema elettorale che lo stesso simpaticissimo collega Calderoli

perché questa è la mia posizione: a mio avviso, l'impegno costituzionale che ciascun parlamentare si è assunto al momento dell'elezione (cioè partecipare all'attività di quest'Aula e determinare, nell'elaborazione e nell'approvazione delle leggi, le regole di vita comune dei nostri concittadini) non può essere messo in discussione da impegni di coalizione o di Governo.

in cui è segnato l'unico vincolo cui ciascuno di noi deve rispondere: quello nei confronti del popolo e dei cittadini che ci hanno eletto a questo altissimo incarico. È questo, per esempio, il limite del metodo attraverso il quale siamo stati eletti in ragione della legge elettorale approvata nell'ultimo scorcio della passata legislatura, che ha eliminato le preferenze, togliendo, quindi, ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio senatore e il proprio deputato. Tale sistema elettorale ha, quindi, indebolito quel «senza vincolo di mandato» scritto a chiare lettere nell'articolo 67 della nostra Costituzione. Ritenendo quel vincolo con gli elettori

Signor Presidente, il dibattito di stasera ha intrecciato questioni di merito a questioni regolamentari;

rispondere ad alcune affermazioni fatte sul diritto al dissenso e sul voto segreto. Mi sembra che proprio la modalità di voto segreto, laddove un senatore non si possa esprimere attraverso l'espressione diretta e palese del voto, debba rendere obbligatoria, come diritto di democrazia, al di là del Regolamento, la possibilità di manifestare la propria opinione. È stato fatto l'esempio della cabina elettorale: ma quando si vota in cabina elettorale (vorrei ricordarlo al senatore Castelli), non c'è un Capogruppo che fa una dichiarazione di voto e che in qualche modo ci impegna; siamo noi, da soli, di fronte all'esercizio di un nostro dovere. Quindi, proprio il voto segreto credo dia a ciascun senatore il diritto di esprimere le proprie opinioni ed il proprio dissenso. Tale dissenso, lo dico garbatamente, dovrebbe avere lo stesso peso dell'assenso; comunque le difficoltà in cui oggi ci dibattiamo in quest'Aula. Vengo alle questioni di merito. Noi abbiamo affrontato più di una volta la questione delle dimissioni dei membri del Governo che intendevano rinunciare alla loro carica di senatori. Abbiamo ricordato anche alcuni precedenti; abbiamo ricordato anche la prassi di cortesia per cui si respingono le dimissioni la prima volta. Ma qui non c'è esclusivamente un problema di democrazia o anche il legittimo confronto rispetto ad un atto che può creare maggiori e più accentuate difficoltà al Governo. Dobbiamo affrontare seriamente la questione dal punto di vista della democrazia e del rispetto del principio di rappresentanza. Ora, vedete, noi abbiamo avuto una legge elettorale prima proporzionale, poi di tipo maggioritario, ora nuovamente proporzionale. Non dobbiamo, con una scelta nostra interna, artare, forzare le scelte degli elettori. elettori. Questa ultima legge elettorale, approvata dal passato Governo e che senz'altro chi mi sta di fronte ben conosce, non consente di fatto all'elettore di esprimere una preferenza e si prefigura effettivamente come una legge elettorale di tipo uninominale, o rientra, più o meno, nello stesso ambito di argomentazioni decisionali. L'elettore che va a votare,

anche territoriale, all'interno dei collegi. Credo, quindi, che il dissenso che oggi esprimo rispetto alle indicazioni date dal mio Gruppo, pur comprendendo le motivazioni di funzionalità del Governo, si sostanzi rispetto a questa analisi che ho tentato di svolgere a proposito del rispetto della rappresentanza. C'è poi un'osservazione che è stata fatta più volte: siamo di fronte ad un voto segreto, quindi molto difficilmente si può dare una riprova.

a rispettare le indicazioni di voto espresse verbalmente con quanto effettivamente si fa nel segreto di questa piccola macchinetta che è davanti a noi. Si può poi - perché succede

un principio di rispetto di noi stessi, dell'Aula e del dibattito che stiamo svolgendo. Vede, Presidente, credo che pacatamente dobbiamo affrontare questa questione. Ho voluto esercitare questo diritto al dissenso perché avremmo

Ma se questo nodo non viene sciolto, a me sembra sia legittimo da parte di ciascuno di noi esercitare quel diritto.

alcune delle questioni che ripetutamente, ormai, sono state sollevate in Aula, concernenti non soltanto i temi odierni, ma anche altre situazioni, per rispetto di noi stessi e dei nostri lavori. Mi verrebbe anche, a questo punto della discussione, abbastanza spontaneo - direbbe un comico - invitare i colleghi senatori a ritirare le loro dimissioni. Non so se poi il Regolamento, non dico il buon senso, lo possa consentire o se è ammesso un ripensamento. Ho la sensazione che in alcuni casi noi senatori, in senso lato, certamente, ma forse non troppo, possiamo anche considerarci una sorta di prigionieri politici dell'Aula. Michiedo anche cosa succederà quando, saremo chiamati a ratificare le decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari rispetto ai seggi contesi, se ci sarà un comportamento un comportamento configurabile come una resistenza da parte dell'Assemblea a far sì che i senatori, democraticamente eletti, non lascino l'Assemblea. dunque un voto di astensione, utilizzando alcuni degli argomenti di chi mi ha preceduto: in particolare, se è vero che nel suo programma in generale l'Unione, e in particolare Prodi, ha ripetutamente cercato di affermare la necessità di distinguere la responsabilità di Governo dalla responsabilità parlamentare, è pur vero che questo problema si pone a tutta la compagine governativa, come ricordava la senatrice

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Bubbico.

i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra.

Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

per favore,

Bubbico cessa di far parte della nostra Assemblea. Rivolgo a lui un apprezzamento e un augurio di buono lavoro altrove.

a meno che, tutti d'accordo, non si proceda alla votazione delle dimissioni del senatore Pinza. Ricordo l'episodio richiamato dal presidente Matteoli e non ho alcuna difficoltà ad accettare la procedura che fissammo l'altra volta, ma qual è il punto,

e ripristinare il *plenum* dell'Assemblea, in sintonia con quanto abbiamo fatto la scorsa settimana. Non vedo perché vi debba essere un comportamento diverso.

credo che il presidente Matteoli abbia ragione in linea di principio, anche se i precedenti

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Basilicata, a seguito delle dimissioni del senatore Filippo Bubbico, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Salvatore Adduce. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Salvatore Adduce. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. Presidenti dei Gruppi si era trovata d'accordo in precedenza sul fatto che la seconda votazione sulle dimissioni del senatore Pinza si svolga nella mattinata di domani.

una nuova finestra"). Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione è convocata

ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge l'ha dichiarata valida: per la Regione Valle d'Aosta il senatore Perrin. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione. Vi comunico, colleghi, la decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo per i lavori di questo scorcio di giornata e per la giornata di domani.

Paolo Ferrero. Dopo le comunicazioni del Governo, seguirà un intervento per Gruppo di dieci minuti ciascuno e non ci sarà nessuna votazione. La seduta terminerà alle ore

Presidente, nella discussione e nei fatti di stamattina sono state poste questioni su piani diversi. Prima di passare alle proposte sul merito, è opportuno

La nostra opinione è che stamattina si sia verificata non una modifica della condizione politica in cui ci troviamo, ma semplicemente una situazione in cui l'assenza giustificata di alcuni senatori della maggioranza ha determinato, in virtù delle determinazioni assunte dall'opposizione, il risultato che conosciamo: non si tratta di una novità, ma di una conferma delle condizioni numeriche in cui ci troviamo al Senato. Dal punto di vista invece del merito della votazione di questa mattina, è evidente che la situazione che ci troviamo a fronteggiare è la seguente. La bocciatura della conversione in legge del decreto del decreto sulgli sfratti determina un doppio problema: il primo è quello dei soggetti deboli che venivano tutelati dal decreto e in particolare dei malati terminali, degli ultrasettantenni, degli invalidi al di sopra del 66 per cento e delle famiglie con minori che, a questo punto, dopo la bocciatura del a fine novembre, di essere coinvolti dalle procedure di sfratto. Il secondo elemento di gravità che deriva dalla bocciatura di questa mattina è che quel decreto conteneva anche la predisposizione di un piano, d'intesa con i Comuni e le Regioni, per ricostruire un intervento sul versante dell'edilizia residenziale pubblica, che era strettamente connessa al blocco degli sfratti. intervento viene a cadere in una situazione che è, come tutti voi sapete, grave su questo versante, non solo

e quello della predisposizione di un piano di edilizia residenziale pubblica), siamo oggi in una condizione di *empasse*. Nel merito sono stati avanzati problemi relativamente alla costituzionalità del decreto. Io voglio sottolineare determinati elementi che poi ci permetteranno di ragionare su come andare avanti. La Corte costituzionale, nel 2004, aveva avanzato alcuni rilievi rispetto al cosiddetto decreto di proroga degli sfratti del 2004 su tre profili: la prima questione, diceva la Corte costituzionale, è che non si può proseguire con mere proroghe degli sfratti. Devo dire che il decreto in discussione questa mattina in Aula era stato costruito in modo da non essere una mera proroga, ma collegava il blocco degli sfratti per le categorie di cittadini particolarmente disagiate ad un piano da costruire con i Comuni e le Regioni; quindi, il rilievo di costituzionalità non poteva toccare questo decreto perché, a differenza dei decreti degli anni precedenti, non prevedeva una mera proroga degli sfratti. senatore Storace)*. Assolutamente no. Il voto è valido e non è contestabile. Sto spiegando le motivazioni sottese al decreto, che porteranno alla proposta che avanzerò alla fine.

che non fosse possibile scaricare sul solo proprietario l'onere di un beneficio sociale più ampio, cioè che non si potesse scaricare sul singolo individuo proprietario che si trovava ad avere in una casa di sua proprietà un inquilino non sottoponibile a sfratto l'onere del medesimo. Per venire incontro

poteva non essere nella condizione di rientrare nel possesso pieno dell'alloggio di sua proprietà perché affittato ad un inquilino malato terminale e, giustamente, la Corte costituzionale segnalava una disparità di trattamento. Anche in questo è stato previsto espressamente che, in caso di parità di condizioni, ci fosse la disponibilità dell'alloggio per il proprietario. Dico questo perché a me pare che il decreto fosse costruito esattamente per rispondere ai nodi di costituzionalità sollevati in precedenza dalla Corte costituzionale. Infine, c'è

in cui non era prevedibile l'esito sulle quotazioni delle società in oggetto. Il Governo sarebbe addivenuto non perché mancasse il finanziamento del decreto, che invece era previsto in altre forme, ma per evitare di intervenire su altre voci del bilancio dello Stato in una modalità non prevedibile, che mi pare fosse uno dei rilievi avanzati della solidarietà sociale*. Chiedo scusa. In questo caso, ho sentito le voci stamattina, nel dibattito cui ho partecipato e a quelle mi riferisco.

sulla precisione del rilievo medesimo. Ciò detto, stiamo verificando con gli uffici

entro la fine di novembre, a risolvere il problema del blocco degli sfratti per queste categorie di persone e a incardinare la costruzione del piano. Per quanto ci riguarda, a partire dalle posizioni dette,

Nel caso in cui le verifiche risultassero negative, evidentemente bisognerebbe passare ad un'ipotesi di disegno di legge. Per quanto ci riguarda, come Governo, così come siamo stati disponibili nel percorso che ci ha portato fino ad oggi, siamo disponibili e interessati a svolgere un dibattito parlamentare - in sede di Commissione o in qualsiasi altra sede si ritenga opportuno

attinenti alla risoluzione del problema in maniera drastica ed efficace. La questione sta nel fatto che il decreto - e quindi il suo Governo, cui lei appartiene

disegno di legge. Mi auguravo che il Ministro, invece di venire a farci - ripeto - la lezioncina sull'importanza di tale decreto, esprimesse anche una considerazione di carattere politico.

in maniera inusitata roboanti, sotto questo profilo, ad un problema molto rilevante, al quale noi, nella scorsa legislatura, in più occasioni abbiamo dato dato risposte, che hanno visto i voti contrari anche della senatrice De Petris, che oggi con tanta cortesia ci ha ricordato la responsabilità che dovrebbe soggiacere all'approvazione di questo decreto. La conclusione è questa: queste belle idee che lei ci ha espresso avranno una maggioranza che permetterà loro di tradursi in un provvedimento legislativo concreto ed efficace? Quello che io chiedo e che la Lega Nord chiede, signor Ministro, è se, dietro alla bocciatura di oggi, ci sia ancora una maggioranza ed un Governo in grado di governare il Paese. Quando si parla, come abbiamo fatto oggi, di responsabilità, mi chiedo: la responsabilità sta in chi

per prendere decisioni drastiche e non si accorge che quindi l'unico che deve essere sfrattato è il presidente del Consiglio Prodi? Sappiamo benissimo che la Costituzione dice che non è un voto contrario ad un provvedimento del Governo, da parte di una o di entrambe le Camere, che ne costringa obbligatoriamente le dimissioni. Non è così, questo è evidente e lo dice anche la Costituzione. Ma non è il primo caso: è successo già sull'ordinamento giudiziario ed in altre occasioni importanti; questa è una di quelle. Non è un caso fortuito o unico. unico. Lei non ci ha dato una risposta; forse non poteva, forse non sapeva, forse, all'interno della collegialità del Governo, non è stata data una risposta e si attendono tempi migliori. È tuttavia gravissima la responsabilità che sta dietro a questo fingere che non ci sia ci sia la questione di una maggioranza che sostiene il Governo, cercando di nasconderla dietro ai valori di un decreto che prorogava gli sfratti e che attuava una miriade di interventi,

e ci dice che in un modo nell'altro cercherà, per amor di patria, di risolvere questo problema o ha bisogno di un Governo che prenda atto che non ha una maggioranza in grado di permettergli di governare in uno dei due rami del Parlamento? Qual è la responsabilità vera? La responsabilità o l'irresponsabilità è quella vostra. È l'irresponsabilità di chi cerca di dimenticarsi (magari grazie anche al fatto che c'è un po' di sciopero in giro nell'informazione), di far passare la nottata, come dicono in certe parti, in modo che domani ci si dimentichi e che, a fronte di qualche altro voto positivo, possa essere superata questa pseudo, finta crisi parlamentare. Non è vero. La realtà dei fatti sta in

punto è la risposta politica che il Governo intende dare al Paese per far fronte gli impegni elettorali che si è assunto, allo scopo, secondo l'illustrazione che ci ha fatto lei anche stasera, di continuare a governare. Questa è la domanda. Lei dovrebbe far capire all'Aula se la politica che intende attuare questo Governo ha un sostegno parlamentare o no. Come? Non lo so. Ce lo dica lei se c'è una maggioranza diversa che può sostenere questo Governo, se d'incanto se d'incanto i parlamentari malati o in missione si ripresenteranno in Aula e saranno sempre presenti; ma sappiamo sia lei che noi che non sarà così. Questa è la risposta che ci attendiamo: e quale altra? Ci dica se lei sarà in grado di approvare un provvedimento in questi termini: senza la fiducia, il decreto fiscale che ci sta arrivando dalla Camera in questi giorni sarà convertito in legge: no! Nonostante le belle intenzioni e le considerazioni di principio, non c'è una risposta a tale quesito. Questo volevo attendere e sapere. Per carità, poteva essere una risposta assolutamente politica e di buone intenzioni; un richiamo alla pseudomaggioranza di centro-sinistra ad essere presente, a votare e ad archiviare quanto successo oggi come un incidente di percorso. di percorso. Spettava a lei, come rappresentante del Governo, venire a riferire in Aula. Invece, non ho sentito nulla sotto questo profilo. Quindi, temo, signor Presidente, che la conduzione politica, la gestione del Governo continuerà facendo orecchie da mercante ai fatti parlamentari che occorrono e che accadono, cercando più o meno di far leva dove sarà possibile in caso di emergenza con il voto di fiducia. Non so quante volte abbiate intenzione di chiederlo. Sempre a questo punto è meglio

ovviamente una assistenza sociale ai provvedimenti del Governo, che voi ritenete così fondamentali. La realtà è questa: non abbiamo avuto risposta al quesito per il quale avevamo chiesto al Governo di presentarsi in Aula. Non abbiamo avuto una risposta univoca, chiara che dovrebbe venire anche dalle altre parti della maggioranza, per chiarire quali sono le politiche che intendete fare a livello parlamentare affinché non succeda quanto successo adesso. Altrimenti, in caso contrario ed opposto, signor Ministro - questo è un messaggio che le voglio adesso comunicare, visto che lei non ci ha dato alcuna indicazione in questo senso - significa che questa è la via della irresponsabilità:

Succederà ancora, signor Ministro, che i decreti verranno bocciati, che i disegni di legge passeranno solo con la fiducia. Quindi, accadrà che il Paese alla fine dovrà pagare in maniera molto cara la irresponsabilità

Signor Presidente, ringrazio ed apprezzo le dichiarazioni del Ministro perché ci riporta tutti - mi dispiace che il richiamo di stamani al senso di responsabilità possa essere frainteso

30 giorni bisogna trovare una soluzione - mi permettodi avanzarne alcune - che venga incontro alla risoluzione del problema. Le pregiudiziali - vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione - non fanno in

abbiamo assistito anche nella scorsa legislatura ad un utilizzo smisurato dei decreti, che non avevano nulla a che fare con l'articolo 77 della Costituzione: non erano cioè certamente basati sui presupposti di necessità ed urgenza. Questo lo era,

una parità tra il locatore e il conduttore (pur sapendo che nel caso delle grandi proprietà tale parità non esiste ma forniva gli strumenti per superare

noi. Capisco che l'opposizione voglia ovviamente tentare strumentalmente di averne un beneficio politico da tutta questa vicenda, però - lo ripeto stasera che siamo tutti più pacati - vorrei invitare ad intervenire e a dare il proprio contributo. Il problema è tutto dinanzi a noi: è nelle città e nella gravità della situazione che si è venuta a creare. Vorrei dire anche con altrettanta

per poter finalmente cominciare in questo Paese, dopo cinque anni in cui il dramma della casa si è solo aggravato, a trovare e a mettere

senatrice De Petris, questo provvedimento non è affatto un buon provvedimento. Siamo purtroppo abituati a vedere le cose dal punto di vista della nostra convenienza politica. C'è un passaggio del programma di Prodi che riguarda l'emergenza abitativa e le sue soluzioni. Ebbene, se la soluzione è quella di questo decreto-legge per fortuna esso non esiste più, grazie a un voto del Senato. È un decreto che mette povera gente contro povera gente; è un decreto non soltanto ingiusto ma dal punto di vista sociale - questo sì - è un mezzo per aizzare le folle. Perché non ci convinciamo una volta per tutte che è vero che esiste un'emergenza abitativa e che delle persone e delle famiglie hanno la necessità del supporto dello Stato? dello Stato, colleghi senatori, non di altri privati; lo Stato costringe, da qualche anno, gruppi di privati a sostenere mancanze di altri gruppi di privati, che noi condividiamo essere mancanze gravi. Come non pensare al pensionato che con lacrime e sangue si è fatto una seconda casetta, o che magari sta in affitto e si è fatto finalmente una casa di proprietà,

stolti e sciocchi ricchi che debbono dare ad altri e, fra questi, alcuni molto furbi e nemmeno poveri. Basta pensare allo scandalo degli IACP. A tal proposito, voglio sapere se il Ministro ha la stessa esperienza dentro che magari hanno fatto gli amministratori locali, anche in grande metropoli come Roma, per esempio. Lo scandalo dello IACP che, quando nacque, grazie alla Democrazia Cristiana,

le vicende della casa e della Democrazia Cristiana, rendendo proprietari in Italia circa l'80 per cento dei cittadini italiani. Ancora molti degli abitanti dei cosiddetti IACP, gli istituti autonomi delle case popolari, sono gli stessi entrati nel 1950, nel 1956, nel 1965, nel 1970. Oggi i loro figli sono affermati dentisti, professionisti, ingegneri, avvocati, ed è giusto che sia così, proprio grazie a quella politica. Sono ancora lì dentro, però, a sottrarre

una dichiarazione di 10.000 euro all'anno per rientrare nella *no tax area* quando invece non sono affatto bisognosi di una casa e stanno alle spalle di un altro privato che magari è bisognoso, dentro il suo appartamento. Si tratta di una legge truffa per questi cittadini italiani che hanno gli stessi diritti di coloro i quali hanno l'esigenza di avere una casa, ma non la loro. Allora, intanto ristabiliamo un principio di equità e di eguaglianza tra i cittadini italiani e finalmente lo facciamo, perché non è il torto di questo Ministro, è una vicenda che si trascina negli anni e in questi governi. Smobilitiamo gli IACP, ad esempio; utilizziamo quei soldi per costruire nuove case per chi veramente ha bisogno, oppure facciamo un buono affitto con quei soldi di 300-400 euro al mese. Liberalizziamo il mercato degli affitti e vedrete come crolleranno i prezzi d'affitto delle case quando stabiliremo con la normativa - ed è una prima proposta che le faccio, Ministro - una cosa non la finita locazione dopo quattro anni, rinnovabili per altri quattro. Tutto passa per anni di cause e qui sono scritte cose - mi scusi se uso questo termine - anche un po' furbescamente, perché si dice che le cause per finita locazione, ma passate in giudicato, sono 12.000. Lei ha idea di quante centinaia di migliaia di cause ci sono per finita locazione che giacciono nei tribunali intasando la giustizia civile - come lei sa bene - e non trovano soluzione da 10-20 anni?

con chiavi in mano al proprietario di casa senza passare per i tribunali e diamo noi una soluzione alternativa. Vedrete come crolla il mercato perché qualunque proprietario di casa, se ha la certezza di rientrare in possesso della propria abitazione dopo quattro o cinque anni, è disponibile anche a diminuire del 30 per cento il valore del contratto di affitto dell'appartamento. Si tratta soltanto di ribadire un principio - e non so se sono tutti d'accordo sul punto - la proprietà privata non è un furto e lo Stato non può approfittare della presunta agiatezza di altri cittadini per risolvere i problemi di chi ritiene essere più povero, ma insisto sulla furbizia di questa fascia. Quanti realmente bisognosi, tra quelli che occupano case di terzi, sono meritevoli di questa attenzione da parte dello Stato?

del Laurentino 38 - e chi conosce questa zona sa che è lo Zen di Roma - ero anche il presidente della squadra di calcio del Laurentino 38 ed ero anche un punto di riferimento in quel quartiere, so bene quali bisogni e quali mancanze vi fossero e da buon democristiano me ne sono sempre occupato: siamo arrivati anche alla demolizione di alcuni ponti, perché totalmente nelle mani della malavita. nelle mani della malavita. Vorrei fare un confronto con Santoro su queste vere informazioni: cosa hanno fatto lo Stato o il Comune per risolvere realmente questo conflitto d'interessi che c'è tra povero e povero? Dobbiamo agire più in profondità, Ministro. Se vuole realmente approfittare dell'occasione, non risolva il problema dicendo «Facciamo un'altra proroga degli sfratti», perché ci saranno migliaia di persone che a queste parole avranno un brivido lungo la schiena, come del resto alcune altre migliaia lo avranno se questa proroga non ci sarà. Allora diamo tempi certi e diamo soluzioni immediate. Quando vedo che si vuole fare un provvedimento del genere senza copertura economica, capisco che non c'è una vera buona fede, perché senza una copertura economica, i Comuni

di tutta l'erba un fascio, perché ci sono Comuni come Rapallo che sono effettivamente Comuni turistici, anche di un certo livello, che secondo questa normativa avrebbero anch'essi case bloccate, magari da qualche furbo.

lei è stato mandato qui - uso un termine che non vuole essere assolutamente offensivo - e come ha affrontato questo suo intervento?

per cui l'Assemblea del Senato ha chiesto la presenza del Governo. Noi abbiamo chiesto la presenza del Governo perché il Governo doveva dimostrare, attraverso il suo intervento, di avere ancora una maggioranza. non è sua competenza specifica, è sua competenza in quanto - mi scusi il bisticcio di parole - è componente di un Governo, ma non è competenza sua. sua. Se affrontiamo l'argomento ed entriamo nel merito, vediamo che in Italia - questo lo diciamo - ci sono stati Governi di centro-sinistra, di centro-destra e centristi, ma non si è mai risolto il problema di fondo su chi deve ricadere il costo dell'abitazione. In Italia, da questo punto di vista, il costo ricade sul proprietario della casa, ricade sull'affittuario quando paga l'affitto o ricade sulla mano pubblica? È un miscuglio che non è mai stato risolto. Ma questo era un argomento da affrontare durante il dibattito sul decreto: un decreto che non c'è più, signor Ministro, perché il Senato l'ha bocciato. iniziando il suo intervento, ha dichiarato (forse le è scappato, mi passi il termine poco parlamentare) che il voto del Senato è grave. Non esistono voti del Senato gravi: i senatori votano liberamente e questa volta hanno votato in un modo diverso da quello che lei auspicava.

Non voglio entrare nel merito del decreto. Il decreto non c'è e non può essere reiterato. L'argomento oggetto della discussione, ripeto, è un altro: siete in condizione di continuare a governare? Se volevate entrare nel merito non del decreto ma del problema

tesa a contattare i *leader* dell'opposizione, oggi maggioranza, per trovare insieme una soluzione. Nessuno vuole, infatti, tanto meno noi, mettere cittadini in mezzo alla strada.

Il problema, ripeto, è politico. Ma non ci sono novità: anche la giornata odierna si è aperta all'insegna della confusione e della contraddittorietà di opinioni all'interno del Governo, tra Governo e maggioranza e all'interno della stessa maggioranza. Ha cominciato questa mattina il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Enrico Letta che, probabilmente per rimediare all'impatto mediatico negativo sulla questione del 45 per per i redditi più alti, è sceso nella sala stampa di Montecitorio per chiarire che il Governo non condivideva l'emendamento presentato dall'Ulivo. Poco dopo, il ministro Damiano (Enrico Letta e Damiano fanno parte dello stesso Governo) in una dichiarazione ha, invece, affermato che l'aliquota del 45 per cento è una buona idea. Per carità, discutiamo pure, ma mettetevi d'accordo: quale delle due strade volete seguire? Successivamente si è proseguito con una ben nota bocciatura del Governo sul decreto sugli sfratti, un

l'Aula del Senato ha battuto il Governo votando una sacrosanta pregiudiziale di incostituzionalità». Ebbene, la maggioranza è stata battuta, in maniera clamorosa, dall'opposizione, divenuta quest'oggi maggioranza,

la colpa è vostra - cioè nostra - se è caduto il decreto che risolveva i problemi abitativi della povera gente. Ma come? Quando vi rivolgete alla destra ci tacciate da padroni della ferriere e ora ci riconoscete una forte sensibilità sociale, tanto che vi meravigliate che abbiamo bocciato il decreto? *(Applausi del senatore

Diceva Lenin che una bugia ripetuta mille volte diventa realtà; ebbene, voi per mille volte avete ripetuto che la destra non si occupava del sociale;

lasciando soli i Presidenti dei Gruppi della maggioranza. Ho apprezzato molto - lo dico senza nessuna ironia, credetemi, perché sono un uomo politico da tanti anni e, quindi,

Avete parlato solo voi perché siete stati lasciati soli dalla vostra maggioranza, dal Governo e dai *leader* di partito, perché non sanno più cosa dire per difendersi, tant'è vero che tant'è vero che il senatore Salvi - come ho detto in un precedente intervento - parla di «una conduzione da parte del Governo che denuncia un agire con un po' di dilettantismo».

tutto si può concedere al presidente del Consiglio Prodi, ma che sia capace di fare ironia è un po' difficile; ebbene, qui ci ha provato e ha detto: «E tutto il resto è musica. Andatelo a dire a Vasco Rossi, non a me». Di fronte a questo, signor Ministro, noi ci aspettavamo una sua presa di posizione nei confronti del Governo per chiarire se avete ancora una maggioranza, se siete nelle condizioni di poter continuare a governare. Il problema del decreto-legge non esiste più: non c'è più, è stato bocciato. Siamo disponibili ad esaminare insieme a voi la possibilità di risolvere il problema degli alloggi, soprattutto per gli aspetti sociali

teso a mettere in evidenza il fatto che il decreto-legge fosse stato bocciato dal Senato, tentando quasi di evitare che si dicesse che ciò è accaduto perché loro hanno votato in un certo modo. Allora, non è una provocazione, non è una provocazione, ma è quasi come se avessero paura che l'opinione pubblica venisse a conoscenza del fatto che questo provvedimento in Senato è stato bocciato perché un certo numero di senatori di una certa parte politica ha votato contro. Io facevo l'avvocato civilista. Se avessi continuato a fare questo lavoro domani avrei preso il «Corriere della Sera» o «Il Sole 24 Ore» e ai clienti che mi avessero chiesto quale fosse la fine dei provvedimenti di sfratto esecutivo e passivo

era uno dei punti nodali, sul quale si sviluppava la discussione e si attagliavano le critiche maggiori dei colleghi dell'opposizione. Probabilmente, staremmo ora discutendo in positivo e non in negativo.

evidenti - dal vostro punto di vista - miglioramenti del testo. Probabilmente in Aula stamattina c'è stata fretta nell'incardinare questioni pregiudiziali e sospensive quando da più parti, non soltanto dalle opposizioni, provenivano richieste di un maggiore approfondimento e di una sospensione.

di aver sbagliato ad impedire che questo provvedimento seguisse il suo *iter* fino alla conclusione, anche attraverso miglioramenti che l'Aula e le Commissioni hanno dimostrato di saper fare.

la recriminazione è che forse era meglio consentire il miglioramento di questo provvedimento in Commissione e poi in Aula, piuttosto che esporci a quella che potrebbe essere - e alcuni lo hanno già fatto - una facile messa in campo di iniziative politiche contro chi, eventualmente, si sia reso artefice di una iniziativa parlamentare che non blocca più gli sfratti dal 29 novembre. Personalmente non farò questo, né lo farà il mio Gruppo politico, però la prossima volta le prove muscolari facciamole su provvedimenti che hanno minore incidenza diretta

nella quale ci siamo riconosciuti in tanti. PONTONE

una di ordine politico generale (e mi auguro che il Ministro possa riferirla al Presidente del Consiglio) e l'altra di ordine più specifico, concernente la questione oggetto del decreto-legge sul quale si è registrato il voto contrario

la prima considerazione di ordine politico: da quando il Governo si è formato, è chiaro che non è possibile governare il Paese avendo in quest'Aula un contesto politico che consente come fatto normale la imprevedibilità di ogni voto su qualunque provvedimento. Questa è la questione politica. Oggi non è un fatto eccezionale il voto contrario a questo decreto-legge, è un fatto del tutto normale. È capitato su questo, poteva capitare ieri, addirittura sull'assestamento di bilancio, su cui il Governo ha avuto la maggioranza perché qualche collega dell'opposizione ha sbagliato a votare, capitare domani su altri provvedimenti importanti. Quindi, la questione politica di fondo, non è il voto contrario di oggi su questo decreto-legge: non è questa l'eccezionalità. L'eccezionalità consiste nel fatto che siamo in presenza di un Governo che afferma di voler governare l'Italia per cinque anni, in un contesto nel quale non ci fa capire come intenda affrontare il problema politico del Senato, non il problema giuridico-parlamentare. Questa è una questione seria.

come il Governo intenda affrontare il problema della governabilità del Paese sulla base del suo programma, sapendo che in ogni momento, su qualunque argomento del suo programma, dal bilancio all'assestamento, alla finanziaria, alle case, alla politica internazionale si corre il rischio di avere una maggioranza che diventa minoranza. Questo è il problema politico. Non dica che si è verificata oggi una situazione eccezionale: oggi è stato colpito, per circostanze fortuite, un pezzo importante della politica del Governo. Ieri poteva essere colpito addirittura l'assestamento di bilancio: lei capisce cosa avrebbe significato questo? Se ieri i nostri colleghi, che hanno sbagliato a votare, avessero votato come avrebbero politicamente dovuto, sarebbe stato bocciato l'assestamento di bilancio e non so con quali conseguenze politiche generali.

è di tutta evidenza che questo programma di Governo, in quanto tale, non è in grado di andare avanti nelle due Camere, soprattutto al Senato, per la imprevedibilità dell'esito delle votazioni,

Detto questo, mantengo il rammarico di non aver avuto neanche un accenno di risposta al riguardo da parte sua e preciso che non ho mai ritenuto che fosse in gioco il Governo in quanto tale oggi; ho ritenuto che oggi fosse accaduto un ulteriore episodio di grande rilievo politico. Non era in discussione questo Governo oggi, ma evidentemente in questo momento il Governo stesso sa di non avere, al Senato, la maggioranza sulle basi fondamentali del suo programma: non su singoli punti, ma su provvedimenti a caso; oggi è capitato sul decreto-legge sugli sfratti, domani può capitare su un'altra cosa. su un'altra cosa. Questo è il problema politico che la giornata del 25 ottobre 2006 pone in evidenza; questo problema non ha ricevuto nessuna risposta e non credo che essa sarà data sabato dall'incontro del vertice cosiddetto di maggioranza del Presidente del Consiglio con i segretari dei partiti che ufficialmente sostengono il Governo se anche lo sostenessero tutti, in modo totale, presenti sempre, non formerebbero la maggioranza strutturale al Senato. Questo è il problema politico che noi abbiamo posto. Vengo alla conseguenza del ragionamento politico:

ho chiesto che il Governo ritirasse il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge che era quello sul quale si era dimostrato lo scontro interno alla maggioranza. È una maggioranza che per un verso ci chiede di approvare un decreto che comporta spese, per un altro verso ci dice che quelle spese non le può sopportare. Questo è il problema di questo Governo: ci sono due filosofie politiche di fondo sul rapporto con la proprietà. Questo riguarda le pensioni, la politica sociale, la finanziaria, la politica estera e quindi anche il decreto di cui lei è sostanzialmente il protagonista principale. Le due filosofie di fondo sull'istituto della proprietà privata sono due filosofie che vengono a scontrarsi in Aula per la semplice ragione che su questo scontro l'opposizione non farà sconti al Governo, è bene che lo capisca. allora la domanda è questa: è in grado il Governo di trovare un punto di equilibrio al suo interno su tale problema, visto che questo decreto‑legge è giunto in Aula con due diverse posizioni, alternative, della maggioranza sul punto fondamentale? Lo risolve questo problema? Dopo ci dirà con quale strumento, disegno di legge, decreto-legge o altro. Comunque, quando avrà risolto il problema interno alla sua maggioranza, risorgerà quello politico generale: su questi temi, con l'opposizione, vuole avere un rapporto preventivo o no? I temi non sono quelli generici di questo o quell'argomento, non sono materie da cosiddetto «inciucio», come ho detto nel mio intervento non si tratta di allargamento della maggioranza o di sostituzione della maggioranza con pezzi da una parte e dall'altra, non c'è nessuna intenzione - parlo come Capogruppo dell'UDC - di fare questo. La domanda è: sulle questioni strutturali questa maggioranza, che è divisa dal punto di vista fondamentale, con l'opposizione si vuole confrontare cercando il punto di intesa, al quale forse faceva riferimento il collega Formisano prima? Formisano prima? Allora potrebbe ottenere una larghissima maggioranza. Lo abbiamo tentato positivamente sul tema della religiosità, pochi giorni fa, approvando all'unanimità una mozione un tema straordinariamente difficile, sul quale non ho motivo di dubitare che la maggioranza abbia opinioni diverse dall'opposizione e all'interno della maggioranza e dell'opposizione ci siano opinioni diverse; ciononostante abbiamo votato all'unanimità.

Ma ovviamente è possibile a una condizione: che la maggioranza ci dica cosa vuol fare della proprietà privata della casa. Deve decidere cosa fare, se cioè ritiene che il proprietario della casa è un delinquente e l'inquilino è una persona per bene, secondo modelli

l'appello al buon cuore nei confronti degli sfrattati, l'ha detto il senatore Cutrufo prima. Occorre capire: siamo in presenza di una politica che vuol far giungere tutti gli italiani alla proprietà dell'immobile destinato alla casa? Allora,

di fare cose che non erano pensabili; in Italia si è giunti a una proprietà privata della casa spaventosa, considerata un bene dal Paese). Se, dunque, il Governo si muove in questo senso, trova il nostro consenso; se si muove contro,

perché nascondersi dietro un dito non serve a nessuno: certamente non serve al Governo, ma non serve neanche a lei. Questo il problema, questo il punto fondamentale: o saltate il fossato, cercando su questo - come su altri punti - un'intesa strategica con l'opposizione,